la questione evidenziata con il presente atto parlamentare verte sul dibattuto tema del mancato adempimento, da parte del datore di lavoro, dell’ordine di reintegrazione del lavoratore disposto dal giudice, in relazione al profilo della effettiva riammissione in azienda e della sua eventuale coercibilità. Al riguardo, secondo l’interpretazione giurisprudenziale prevalente, la condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato ha ad oggetto un facere infungibile e come tale non può essere coattivamente eseguita. Secondo il costante orientamento della suprema Corte in materia di reintegra, risulta indispensabile e insostituibile un comportamento attivo da parte del datore di lavoro consistente nell’impartire al dipendente le opportune direttive e le misure atte a ripristinare una relazione di reciproca e infungibile collaborazione. Diversamente, il reinserimento del lavoratore nel libro paga o matricola, il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e il pagamento delle retribuzioni rientrano tra le prestazioni cosiddette fungibili, che sono invece suscettibili di esecuzione coattiva. Tanto premesso, con riferimento alla vicenda in esame, il Ministero della giustizia ha reso noto che il 14 marzo 2017 il giudice del lavoro presso il tribunale di Gorizia ha pronunziato quattro ordinanze, tutte di analogo contenuto e immediatamente esecutive. Con tali ordinanze, il giudice del lavoro ha accolto i ricorsi proposti da quattro lavoratori avverso i licenziamenti intimati nei loro confronti da Fincantieri SpA, disponendo la loro reintegrazione, unitamente al pagamento delle retribuzioni maturate medio tempore, alla ricostituzione delle posizioni previdenziali assicurative e alla rifusione delle spese di lite. Avverso le predette ordinanze, lo scorso 13 aprile, la Fincantieri SpA ha proposto ricorso per opposizione, legge 28 giugno 2012, n. 92, innanzi al tribunale di Gorizia. Martedì 25 luglio il giudice del lavoro ha pronunziato quattro sentenze, tutte di analogo contenuto, con le quali ha rigettato tali opposizioni, accertando l’illegittimità della sanzione disciplinare espulsiva e disponendo altresì la reintegra immediata dei lavoratori. Fincantieri SpA è stata inoltre condannata a ricostituire la posizione assicurativa e contributiva dei lavoratori, nonché a corrispondere ai medesimi la retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra effettiva, entro il limite di dodici mensilità. Infine, occorre evidenziare che nel caso in esame, essendo intervenuti i licenziamenti nella vigenza del vecchio regime di cui all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, i lavoratori licenziati possono chiedere, in luogo della reintegra, un’indennità sostitutiva pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto.

la copertura degli aspetti assicurativi e assistenziali; altra cosa è entrare effettivamente nel posto di lavoro, cosa che non era stata consentita. Sembra paradossale e incredibile, ma lo stipendio percepito rispondeva una prestazione lavorativa non erogata. Questo aspetto sembra essersi assolutamente risolto e sono assolutamente soddisfatta

con l’atto di sindacato ispettivo in trattazione, il senatore interrogante, dopo aver svolto una sintetica esposizione di alcuni passi della testimonianza resa dal presidente

sul tenore delle dichiarazioni predette e sulla documentazione trasmessa dall’Autorità medesima alla procura della Repubblica di Roma, richiede al Ministro di sapere se sia a conoscenza della vicenda, se ne sia stata valutata l’incidenza sull’andamento dell’attività giudiziaria e sullo specifico processo e se questo Ministero intenda assumere iniziative ispettive per appurare eventuali irregolarità connesse alla vicenda. Come è noto, il processo in parola è stato definito in primo grado con sentenza del tribunale di Roma del 20 luglio. Esula, ovviamente, dalle prerogative del Ministro della giustizia esprimere valutazioni di qualsiasi natura sulla decisione, della quale peraltro si conosce il solo dispositivo, e per di più in ordine alla rilevanza e incidenza di una testimonianza sul libero convincimento dei giudici. La vicenda, tuttavia, è stata compiutamente e autonomamente tratteggiata dal presidente dell’Autorità anticorruzione, in una missiva diretta al Ministero della giustizia, nei termini che seguono. In data 22 dicembre 2014, dopo che la stampa aveva dato notizia dell’indagine svolta dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, l’Autorità nazionale anticorruzione ha ritenuto di trasmettere all’autorità giudiziaria un primo resoconto delle verifiche già disposte, per appurare se fossero stati effettuati in passato degli specifici accertamenti sugli appalti relativi ai servizi sociali; unitamente al resoconto, veniva trasmessa alla procura la documentazione rinvenuta agli atti dell’Autorità. Secondo quanto riferito, sarebbe emerso che negli anni 2010-2011, l’Autorità (all’epoca denominata Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) aveva posto in essere effettivamente attività ispettive nei confronti del Comune di Roma, all’esito delle quali era emersa una serie di criticità connesse alla gestione di strutture da adibire all’accoglienza dei cittadini immigrati. Nella seduta del 20 luglio 2011, l’Autorità aveva ritenuto di non adottare un provvedimento riferito alla sola Roma Capitale, ma di procedere a una comparazione tra le descritte modalità di gestione con quelle adottate in altre città, effettuando ulteriori indagini ispettive. Nella nota trasmessa il 22 dicembre 2014 alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, si osservava che «nessuna attività di successiva ispezione è stata effettuata né in alcun modo è stata effettuata comparazione con altre città né che le irregolarità comunque emerse, siano state comunicate al comune di Roma o rese note alla Corte dei Conti o alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma”; Una volta svolti ulteriori approfondimenti, in data 8 ottobre 2015 l’Autorità dava comunicazione alla procura della Repubblica che dalle verifiche effettuate non era emerso un quadro sostanzialmente diverso da quanto già reso noto il 22 dicembre 2014; per mera completezza, veniva trasmessa alla stessa procura ulteriore documentazione rinvenuta agli atti. Quanto ai rilievi mossi nel corpo dell’interrogazione, il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione osserva che, contrariamente a quanto ipotizzato nell’atto di sindacato ispettivo, alcuna comparazione tra la gestione di Roma Capitale e la situazione rilevata presso altri Comuni è stata mai effettivamente svolta: stando a quanto osservato, la delibera n. 25 datata 8 marzo 2012, infatti, «si riferisce esclusivamente ai Comuni di Bari, Bologna, Foggia e Torino» e nella stessa, salvo un riferimento generico alla situazione di Roma Capitale, «non vi è traccia di alcuna comparazione tra le attività poste in essere dal Comune di Roma e i quattro Comuni ispezionati». Stando alla ricostruzione offerta, a differenza di quelli citati, il Comune di Roma «non è stato oggetto di alcuna specifica delibera, né di specifiche raccomandazioni in merito alle criticità rilevate a suo tempo dall’ufficio». Sulla specifica vicenda, attraverso la competente articolazione ministeriale, sono state richieste informazioni all’autorità giudiziaria. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che «il dottor Raffaele Cantone ha trasmesso, in data 22 dicembre 2014, una nota in cui veniva prospettata l’ipotesi di possibili irregolarità nell’attività svolta negli anni precedenti da parte di dipendenti dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici in relazione ad alcuni appalti affidati dal Comune di Roma a società cooperative». Il procedimento iscritto in base alla predetta relazione - ha riferito il procuratore - è stato successivamente archiviato. Un ulteriore profilo di criticità segnalato dal senatore interrogante sull’operato dell’Autorità nazionale anticorruzione nella vicenda riguarderebbe un documento allegato alla nota del 22 dicembre 2014: si tratta di copia della relazione «Appalti di servizi sociali da parte di Roma Capitale, fascicolo GE/10/73444», in cui non comparirebbe più, come nell’originale, la firma del direttore generale che l’aveva trasmessa il 6 luglio 2011 al consiglio dell’Autorità. Quanto alla rilevanza penale della difformità cui allude l’interrogazione, esula dalle attribuzioni del Ministro ogni valutazione in merito, essendo evidentemente rimessa la questione all’autorità giudiziaria. Si riportano, tuttavia, le valutazioni offerte al riguardo del presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione sull’episodio. Secondo la ricostruzione offerta, la relazione «Appalti di servizi sociali da parte di Roma Capitale, fascicolo GE/10/73444», trasmessa alla procura della Repubblica il 22 dicembre 2014, è quella firmata dal dirigente e dal funzionario istruttore, regolarmente protocollata in data 6 luglio 2011. La stessa relazione è stata per completezza allegata anche alla già citata nota dell’8 ottobre 2015, diretta ancora alla procura della Repubblica di Roma. Prosegue la nota dell’Autorità anticorruzione: «Anche se le due relazioni sono perfettamente speculari nel contenuto, la seconda è priva del protocollo e reca il visto del dirigente generale competente». Con la nota medesima viene offerta una spiegazione dell’episodio nei termini seguenti: «La predetta discrasia appare facilmente comprensibile conoscendo gli strumenti interni e le modalità di lavoro. Infatti, posto che il contenuto delle due note è perfettamente identico, sembra possibile presumere che il direttore generale abbia apposto il proprio visto sulla relazione quando ancora non era stato riportato sul documento originale l’etichetta con il numero di protocollo già acquisito mediante il sistema informatico. Il funzionario competente, infatti, una volta protocollato il documento - rimane agli atti dell’Autorità in formato elettronico ed è quindi immodificabile - deve riportare sul documento originale il corrispondente numero protocollo. Ciò può essere effettuato o stampando l’etichetta o riscrivendo materialmente il numero sul documento. È possibile presumere, pertanto, che il visto del direttore generale sia stato apposto quando materialmente il numero di protocollo non era ancora stato trascritto sul documento originale. Tale ipotesi trova conforto anche nelle dichiarazioni che lo stesso direttore generale ha effettuato dinanzi alla commissione ispettiva interna; questi ha, infatti, dichiarato di aver apposto il proprio visto in data 8 luglio 2011, mentre il documento risulta protocollato il 6 luglio 2011». Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che, a seguito di quanto prospettato nell’interrogazione, è stato iscritto un procedimento a modello 45, allo stato pendente. L’intera vicenda, dunque, risulta al vaglio dell’autorità giudiziaria sia con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni rese in sede di testimonianza dal presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, sia per quanto attiene alla discrasia documentale cui si è fatto cenno. In questa fase, quindi, non appaiono ricorrere i presupposti per alcun tipo di intervento da parte del Ministero.

la risposta che ovviamente non mi trova del tutto soddisfatto anche perché il processo ex Mafia Capitale c’è stato, abbiamo visto com’è andato a finire e ovviamente è venuto fuori che c’era un vero sistema

l’interrogante guardava alle deposizioni rese in quel processo. Poi la Sottosegretaria ha detto che circolano documenti, con firma o senza firma,

Capitale con cooperative sociali, predisposta dalla direzione vigilanza, lavori, servizi e forniture della prima, ne aveva rinviato l’esame senza eseguire alcuna successiva attività di ispezione o di comparazione con altre città o contestato alcunché in ordine alle illegittimità ivi rilevate. Tuttavia, in quella deposizione è stato dimenticato di riferire - perché io non l’ho trovato, ha detto adesso la Sottosegretaria e mi sarebbe piaciuto vederlo in quel processo, in quella deposizione - sia alla procura sia nella testimonianza al processo, che con la delibera n. 25 del 2012, pubblicata sul sito, l’Autorità di vigilanza aveva viceversa concluso l’indagine sugli appalti pubblici delle cooperative sociali con contestazioni ai Comuni presi in esame tra i quali Roma Capitale.

185 del 2012, che la Sottosegretaria può consultare, l’Autorità aveva emanato le opportune linee guida in materia, raccomandando il ricorso a bandi e gare nel rispetto della concorrenza e del codice dei contratti e ciò nonostante il legislatore, con con la legge n. 135 del 2012, avesse poi inteso sanare quelle stesse illegittimità formulando addirittura apposite deroghe anche per l’avvenire. Quindi, noi le abbiamo sanate ma prima c’erano.

dalla stessa Autorità, dalla stessa presidenza alla procura, la relazione del 20 luglio 2011, pubblicata dal sito web del giornale «Il Fatto Quotidiano» il 15 settembre 2015, e che si può scaricare, risultava cancellata la firma del dirigente generale che aveva proposto inizialmente di rinviare l’indagine sulle cooperative sociali. Non era mancante, era cancellata. Firma che, viceversa, compariva nell’originale trasmesso ai consiglieri dell’Autorità.

o distrattamente non riferite. È per questo che abbiamo chiesto al Ministero se era opportuno

Sono state dette cose che si potevano non dire. Quello che invece si doveva dire e che era necessario dire non si è detto. Non si può qui affermare: manca una firma.

non è soddisfatta la legalità, perché riteniamo che forse non c’è alcun reato, ma volevamo sapere perché circolano alcuni documenti con firma e altri senza firma, perché si danno alcuni documenti e non se ne danno altri. Forse per distrazione, forse perché invecchiando tutti quanti perdiamo memoria: anche questa è una spiegazione. PRESIDENTE.

ordine del giorno: I. Discussione del disegno di legge: Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Approvato dalla Came_ra dei deputati; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla_ Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale) - Relatori MARINO Luigi e TOMASELLI